L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Colleghi, non ho intenzione di alzare la voce oltre questo livello per coprire il brusìo e la confusione che ci sono in Aula. Se continua così, applico la regola del presidente Schifani e sospendo la seduta per cinque minuti.

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sul disegno di legge n. 1306 di conversione del decreto‑legge 30 dicembre 2008, n. 208, i lavori della Commissione sono stati caratterizzati dall'aperto e appassionato confronto fra tutti i Gruppi parlamentari e da un ricco e approfondito dibattito, al quale hanno fornito un rilevante contributo tutti i componenti della Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che ringrazio sin d'ora, e il rappresentante del Governo, il sottosegretario Menia. Questo confronto ha avuto come esito, da una parte, la conferma delle scelte normative recate dal provvedimento, ad alcuni profili delle quali la Commissione ha peraltro ritenuto di dover conferire una maggiore precisione e una più puntuale configurazione, attraverso l'approvazione di alcune proposte emendative ora sottoposte all'Assemblea. Dall'altra parte, la Commissione ha ritenuto necessario approvare una serie di emendamenti di carattere aggiuntivo, finalizzati ad inserire nel provvedimento disposizioni volte in particolare a rafforzare l'azione delle pubbliche autorità a salvaguardia dell'ambiente, a promuovere iniziative e progetti di educazione ambientale nella scuola superiore e nelle università, a valorizzare il mercato dell'usato nella prospettiva fondamentale della prevenzione e riduzione dei rifiuti, ad agevolare la realizzazione di interventi di recupero ambientale di siti, in particolare seguendo indirizzi già espressi dalla Commissione al termine di sue indagini conoscitive effettuate in questi mesi riguardo ad alcuni specifici settori produttivi. All'articolo 1 del decreto in conversione, si novellano le norme transitorie relative all'autorità di bacino, contenute nell'articolo 170 del codice ambientale al fine di prorogare le stesse autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 63, comma 2, dello stesso codice ambientale. L'articolo 2 del decreto-legge introduce una forma di risoluzione stragiudiziale del contenzioso relativo alle procedure di rimborso delle spese di bonifica e ripristino di aree contaminate e al risarcimento del danno ambientale.

Si tratta di una innovazione normativa finalizzata a segnare un salto di qualità rispetto all'attuale situazione, caratterizzata dal frequentissimo e spesso inconcludente contenzioso che sorge in riferimento alle stesse procedure per il rimborso. Del resto, Del resto, l'istituzione di una procedura alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie appare capace anche di consentire un recupero in tempi certi delle aree contaminate. L'articolo 3 reca una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in particolare in considerazione del fatto che almeno un terzo delle attività istituzionali è attualmente assicurato attraverso l'impiego di personale non legato all'Istituto da un contratto di lavoro a tempo indeterminato; per questo motivo, in assenza di un intervento legislativo, interi settori di intervento sarebbero posti a rischio

l'articolo 4 del decreto prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze apporti con propri decreti, e su proposta del Ministro per l'ambiente, le variazioni in bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base,

della legge n. 244 del 2007 e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e renderebbe più agevole e rapida l'efficacia e l'operatività della stessa Commissione. L'articolo 5 del decreto modifica le disposizioni legislative vigenti allo scopo di prorogare a tutto il 2009 il regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in attesa della definitiva adozione degli atti necessari all'implementazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani introdotta dall'articolo 238 del codice dell'ambiente. A seguito della nuova proroga, i Comuni dove nel 2006 vigeva ancora la TARSU continueranno ad applicare anche nel 2009 la tassazione prevista dal decreto legislativo n. 507 del 1993, mentre gli enti che nel 2006 avevano già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal decreto legislativo n. 22 del 1997 dovranno continuare ad applicare tale tipologia di entrata.

La Commissione è entrata nel merito della proposta governativa e ha apportato importanti modifiche che affronteremo nel corso dell'esame degli emendamenti approvati in Commissione. L'articolo 6 del decreto in conversione proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti che presentano

con il quale è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Tale divieto, non previsto dalla direttiva comunitaria, era stato inserito nel decreto legislativo n. con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione. L'articolo 7 interviene sulla normativa che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'articolo 8 prevede il finanziamento della spesa di 100 milioni di euro per fronteggiare le situazioni di emergenza a seguito dei fenomeni alluvionali verificatisi nel mese di dicembre. Le risorse dovranno essere ripartite con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i commissari all'emergenza sono chiamati a rendicontare la loro attività entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio. La Commissione ha approvato alcuni emendamenti volti ad introdurre anche commi aggiuntivi all'articolo 8, in particolare al fine di stanziare 19 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008 in Emilia Romagna, nonché al fine di consentire l'applicazione anche alla componente volontaristica della Croce Rossa e ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, impiegati in attività di protezione civile, della disciplina relativa alla partecipazione a queste attività delle organizzazioni di volontariato. La Commissione ha approvato, inoltre, alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 al fine di favorire l'utilizzo di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione di marmi e pietre per interventi di miglioramento ambientale di siti e per interventi di recupero ambientale, nonché al fine di disciplinare compiutamente le modalità di utilizzo e collocazione dei materiali dì risulta di attività di dragaggio e pulitura dei porti. La Commissione, infine, ha approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a dare concreta attuazione al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette», sottoscritto in data 1° febbraio 2007; a predisporre i decreti istitutivi e i regolamenti per tutte le aree marine protette in coerenza con i contenuti del Protocollo tecnico; ad adottare rapidamente i nuovi regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto ecocompatibili; ad indicare le ulteriori misure di premialità per gli scafi a basso o nullo impatto, riconoscendo la propulsione ibrida al pari di quella elettrica quando utilizzata in modalità «emissioni zero»; ad avviare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera. La Commissione infine - e questo è un punto assai rilevante, Presidente, colleghi - ha, altresì, dibattuto il tema dei rimborsi agli utenti per il servizio di depurazione non effettuato nell'ambito dei più complessi servizi idrici. Ricordo che il diritto al rimborso è stato sancito dalla Corte costituzionale con sentenza dell'ottobre 2008 e che moltissime procedure sono state congiuntamente già avviate in tutto il territorio nazionale ai fini di ottenere lo stesso rimborso. Nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale ed a seguito degli approfondimenti scaturiti dal dibattito in Commissione, nella qualità di relatore ho depositato un testo di applicazione della sentenza che salvaguarda il diritto al risarcimento nella condivisione del principio che i corrispettivi dei servizi, non essendo tributi, non sono dovuti quando il servizio non è reso, e che altresì disciplina il rimborso, la definizione del *quantum* e le modalità di corresponsione riportandole ad un - spero condiviso - criterio di ragionevolezza e di contenimento Signor Presidente, come i colleghi potranno rilevare da una attenta lettura anche delle proposte emendative nei lavori svolti in Commissione vi è grande attenzione per le tematiche ambientali, da parte del Parlamento come, peraltro, da parte del Paese e del Governo. In particolare, la Commissione ha ritenuto di dover intervenire su alcune modifiche al cosiddetto codice ambientale del 2006, in più parti variato dal precedente Governo nel 2008. le modifiche proposte, dopo il saggio filtro del quale ringrazio i componenti tutti della Commissione ed il rappresentante del Governo che ne ha puntualmente seguito i lavori, sono certamente una piccola parte di quelle che erano state presentate e di quelle contenute quelle contenute in numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati al Senato. Ciò è significativo - ripeto - della volontà del Parlamento che interpreta la volontà del Paese, così come è chiara la volontà di recepire importanti direttive comunitarie, prima tra le quali la n. 98 del 2008 in materia di riclassificazione dei rifiuti e delle materie prime-secondarie. Sono argomenti, le modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 e le modifiche a numerose leggi in materia di salvaguardia dell'ambiente ormai datate da oltre quindici anni, che nei prossimi mesi, ove dovessero non intervenire le attese proposte governative, la Commissione non esiterà ad affrontare. È stato È stato da più parti ed in più parti giustamente affermato che una corretta e costruttiva politica ambientale può utilmente contribuire anche al superamento della crisi economica in atto. Noi ne siamo convinti ed auspichiamo di poterne presto discutere i contenuti.

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento che discutiamo oggi è una sorta di *omnibus* ambientale, affronta molti temi e quasi sempre si tratta di temi di grande rilevanza. In molti casi, la necessità e l'urgenza di un intervento legislativo è pienamente condivisibile, ma la direzione delle soluzioni proposte riteniamo sia spesso lontana da quelle stesse necessità ed urgenza. E come ormai d'abitudine per questo Governo e questa maggioranza nel decreto sono state introdotte norme che di necessario e di urgente hanno solo l'obiettivo di rafforzare, talvolta impropriamente, il controllo dell'Esecutivo su scelte, su politiche, squisitamente di competenza delle Regioni o di procedere ad una parziale ma rilevante riscrittura della legislazione ambientale, che certamente non può rivestire la forma del decreto-legge. In Commissione ambiente abbiamo svolto una discussione approfondita e non formale sul decreto n. 208 all'esame, e di questo do atto volentieri al presidente D'Ali, che del decreto è anche relatore. Alcuni suggerimenti del nostro Gruppo sono stati accolti, ma restano da parte nostra notevoli perplessità sull'impianto e sui contenuti di questo testo. Comincio dagli articoli l e 2, forse quelli di più vasta e generale portata. L'articolo l si occupa della fase transitoria verso l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, quali previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006; lo fa cancellando, in particolare per i distretti idrografici in cui sono presenti autorità di bacino di rilievo nazionale (che poi sono quelli più importanti), ogni ogni ruolo delle Regioni e delle altre autorità territoriali con competenze in materia di difesa del suolo e di governo del ciclo delle acque. un emendamento presentato dal relatore interviene sulla sentenza della Corte costituzionale che ha disposto la restituzione agli utenti delle somme pagate per i servizi di depurazione nei casi in cui non vi siano i depuratori. Il principio fissato dalla Corte è naturalmente condivisibile. La norma proposta demanda al Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e dei parametri di tali procedure di restituzione. Per quanto ci riguarda, crediamo indispensabile che tale definizione risponda a due esigenze irrinunciabili (e sulla base della misura in cui tali esigenze verranno accolte nelle decisioni del Ministro valuteremo anche il nostro giudizio). Tali esigenze sono, in primo luogo, quella di salvaguardare le situazioni in cui i depuratori, sebbene non ancora funzionanti, siano finanziati o addirittura in costruzione, luogo, quella di determinare un meccanismo di compensazione ambientale tale per cui sia adeguatamente contabilizzato anche nella tariffa, nelle forme che si riterranno più idonee, il danno ambientale prodotto dagli scarichi non depurati. Insomma, è vero che chi ha pagato un servizio non reso va rimborsato, come ha stabilito la Corte costituzionale, ma è altrettanto vero che chi scarica nei corpi ricettori reflui non depurati deve essere chiamato, sulla base del principio "chi inquina paga", a risarcire il danno che ne consegue. L'articolo 2 del decreto affronta un altro tema di grande rilievo, legato all'esigenza di definire i contenziosi in atto per ciò che riguarda il risarcimento del danno ambientale nei siti inquinati d'interesse nazionale. Anche in questo caso l'impostazione del testo rivela un carattere marcatamente centralistico. La soluzione prospettata affida infatti al Ministero il compito di stabilire i termini di una transazione con le imprese chiamate a risarcire il danno attraverso lo strumento della conferenza di servizi. Il contratto transattivo ha l'effetto di porre fine ad ogni contenzioso pendente, ma poiché non è chiarito se e come tutti gli enti territoriali coinvolti partecipino alla decisione il rischio concreto è l'estromissione degli stessi dalla reale partecipazione all'assunzione delle determinazioni che li riguardano. In parole povere, la fine del contenzioso riguarderebbe anche enti che non hanno aderito al contratto, ledendone con ciò il diritto alla difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. Dell'articolo 5, che riguarda il tema dei rifiuti, parlerà più diffusamente la collega Mazzuconi, io mi limito a ricordare che in questo caso l'accoglimento di proposte avanzate dal nostro Gruppo ha consentito di modificare il testo evitando che per tutto il 2009 fosse necessariamente impedita per i Comuni la possibilità di passare, per ciò che riguarda la forma di pagamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dal sistema della tassa a quello, assai più equo e razionale, della tariffa. L'articolo 8, recante disposizioni in materia di protezione civile, è fondamentalmente una grande occasione perduta. Su questo dirà meglio di me la senatrice Soliani. A me preme sottolineare che di fronte al ripetersi, sistematico ahimè, di eventi che dimostrano la necessità di un forte impegno, anche in termini finanziari, per fronteggiare gli effetti di singoli eventi calamitosi (penso al terremoto che ha colpito nel dicembre scorso le province di Modena e Reggio Emilia o alle frane che hanno devastato vasti territori della Calabria e non solo), di fronte all'allarme lanciato ripetutamente dal capo della Protezione civile Bertolaso, che, anche intervenendo nella nostra Commissione, ha lamentato i tagli portati dal Governo alle spese per la difesa del suolo e per la Protezione civile, di fronte a tutto ciò, Governo e maggioranza si sono dimostrati pressoché indisponibili a prendere atto di un dato di banale e drammatica evidenza. Il dato è quello del dissesto e della fragilità del territorio italiano: il 77 per cento dei Comuni italiani dichiara di avere una parte del proprio costruito in aree a rischio. tratta di un grande problema nazionale, che comporta costi elevati in termini di sicurezza e spesso anche di vita dei cittadini, di tutela ambientale ed anche in termini economici. il Governo ha dimezzato gli stanziamenti per la difesa del suolo, portandoli da 540 a 270 milioni, ed ha azzerato il fondo regionale della Protezione civile. Il decreto-legge n. 208 poteva essere, ma finora non è stato, l'occasione per porre un primo, sia pur parziale, rimedio a questo gravissimo errore. Infine, mi fermo brevemente su due dei tanti emendamenti aggiunti dal Governo e dal relatore in dirittura di arrivo: quelli che istituiscono la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche e l'Unità tecnica sui rifiuti. L'obiettivo di tali norme, anche in questo caso, è di banalissima evidenza: cambiare nome al COVIRI (Comitato di vigilanza sulle risorse idriche) e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, organismi già esistenti e pienamente operativi, con il solo scopo di poterne rinominare componenti e vertici. Si tratta pertanto di uno *spoils system* all'amatriciana, lo stesso già utilizzato dal Governo e, in particolare, dal Ministero dell'ambiente nel caso dell'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio), delle Commissioni per la valutazione ambientale, dell'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica). In particolare, nel caso del COVIRI, l'esito di questa misura è di preludere all'allontanamento di un tecnico di indiscusso valore come il professor Passino, che attualmente lo presiede e che certamente non è considerabile un uomo di parte. La scelta è resa ancora più contestabile dal fatto che alla nuova - si fa per dire - Commissione viene affidata, tra l'altro, la «predisposizione del metodo tariffario per la determinazione della tariffa idrica»: non la definizione delle componenti di tale tariffa, che in effetti spetta all'autorità centrale, ma la determinazione della tariffa che invece è di competenza delle Regioni. Ripeto e concludo. Il PD in Commissione ha fatto ogni sforzo per collaborare con la maggioranza al miglioramento del decreto-legge in esame. In qualche caso ci siamo riusciti; in molti altri, invece, alla disponibilità della maggioranza ha fatto da contraltare la chiusura del Governo, che ha costretto a trasformare diversi emendamenti largamente condivisi in ordini del giorno. Alla fine - questo è per ora il nostro giudizio - il testo che arriva in Aula ci appare complessivamente insoddisfacente.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame si occupa di materia varia e diversa ed è stato ulteriormente implementato da emendamenti del Governo e del relatore. La materia è dunque - lo ripeto - assolutamente varia e non riconducibile a sintesi. perciò soffermarmi solo su alcune questioni che ritengo fondamentali, legate l'una all'articolo 5 del decreto-legge, l'altra un emendamento del Governo in materia di valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato tendente ad Nel primo caso - mi riferisco all'articolo 5 - la previsione di prorogare ulteriormente il blocco della TARSU, che è in vigore nella maggiore parte dei Comuni, e della TIA per una minoranza di Comuni,

Perché il Ministro dell'ambiente non adempie al dettato dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prescriveva, già parecchi mesi or sono, la stesura di un regolamento in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani? Perché non vengono dati i criteri generali sulla base dei quali definire le componenti dei costi e dunque il metodo della tariffa stessa, nonché le eventuali agevolazioni che potrebbero riguardare, ad esempio, le zone rurali e le famiglie numerose? Perché questa esitazione? Perché non passare alla tariffa, legando alla stessa una previsione premiale per chi produce meno rifiuti rispetto alla media nazionale e per quelle azioni positive dei cittadini, degli enti locali e dei loro enti strumentali, che concorrano a diminuire la produzione dei rifiuti? Parliamo tanto di diminuzione dei rifiuti, ma non si fa mai nulla perché si diminuisca detta produzione. Si parla molto della raccolta differenziata, meno di questo elemento altrettanto importante. Orbene, la tariffa sarebbe un utile strumento in tal senso; non solo, molti Comuni virtuosi si erano già preparati al passaggio da TARSU a TIA, avevano disposto studi, interventi e modifiche dei sistemi informatici, ma sono rimasti bloccati dopo avere investito cospicue risorse, da una norma che ormai da 2 anni impone, non si comprende con quale criterio, che i Comuni che applicano la TARSU continuino obbligatoriamente ad applicarla, così come, ovviamente, quelli che prevede l'articolo 5 del decreto che dispone una ulteriore proroga della materia, un ulteriore blocco. Si comprendono le difficoltà per alcuni Comuni, soprattutto quelli in emergenza ambientale, a passare dalla TARSU alla TIA, non c'è chi non veda

Che cosa impedisce oggi ai Comuni di individuare aree per lo svolgimento periodico di mercati dell'usato? Praticamente nulla e nessuno, eppure abbiamo questa previsione inserita con un emendamento del Governo. invece una questione seria per le aree che hanno raggiunto elevati livelli di raccolta differenziata perché non è in alcun modo consentita la commercializzazione di beni usati e funzionanti, raccolti nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti. Ad essi viene tassativamente applicato, in ingresso agli impianti, un codice del catalogo europeo dei rifiuti, il cosiddetto codice CER, e non è possibile procedere alla vendita di tali beni. Dunque tali materiali non potranno concorrere alla riduzione dei rifiuti

delle tariffe e del costo della vita. Senza contare che in questo campo abbiamo un importante apporto da parte dei soggetti *non profit* che, ovviamente, sono i primi a riutilizzare questa materia anche a fini sociali e non solo per la vendita. Ovviamente tutto questo andrebbe svolto presso impianti autorizzati e con regole precise, e potrebbe essere supportato da autorizzazioni provinciali opportunamente modificate per quanto riguarda le piattaforme ecologiche e comunque gli impianti di smistamento, ma nulla di ciò è presente, né nel decreto, né nell'emendamento aggiuntivo del Governo. Il Gruppo del PD ha presentato dei subemendamenti che speriamo vengano accolti. Molti poi sono gli argomenti introdotti dagli emendamenti del Governo, che però non si occupa di vicende importanti come, ad esempio, quelle legate ai gravi eventi alluvionali che hanno colpito recentemente il nostro Paese, e segnatamente la Calabria. Già in altre occasioni - lo ricordava prima il collega Della Seta - il sottosegretario Bertolaso, in Commissione ambiente, ha chiesto risorse e lamentato il taglio di risorse avvenuto nelle varie sedi. Ma dove sono queste risorse?

Dissesto idrogeologico, protezione ambientale, protezione civile non ricevono mai l'attenzione che meriterebbero in questo momento storico della vicenda italiana. Lo avevamo già detto in sede di esame del DPEF e lo ribadiamo ora

Non è corretto però che le questioni compaiono sempre a pezzi e mai in un quadro complessivo. Prima parlavo della protezione civile, del dissesto idrogeologico e della protezione ambientale in genere,

che davvero non fanno ben sperare. Torniamo anche alla questione della gestione del ciclo integrato. Abbiamo bisogno di un quadro certo, definitivo e duraturo nel tempo:

altrimenti, anziché andare verso la soluzione dei problemi, andremo sempre di più verso la confusione, il cattivo servizio a danno dei cittadini, il danno ambientale,

Mazzuconi. Già allora demmo una delega in bianco al Governo e si parlava di provvisorietà; dissi allora che non c'è niente di più definitivo che il provvisorio nel nostro Paese. Oggi ancora proroghiamo la possibilità di portare in discarica l'indifferenziato fino al 31 dicembre 2009. Questo non dico che serva ad incentivare i Comuni a non farlo, ma serve a non dare una mano ai Comuni ad imporre la raccolta differenziata. Già abbiamo questo problema in Campania; è stato un evento nazionale. Vi abbiamo detto che

non possiamo farveli passare, anche perché tutte queste proroghe sono un danno per l'amministrazione dello Stato.

Con questo decreto il Governo adotta numerose proroghe in materia ambientale ed introduce una disciplina ulteriore in materia di danno ambientale. Va preliminarmente osservato come la pratica, in verità non nuova ma ormai sistematica, dell'adozione di provvedimenti legislativi di proroga di disposizioni vigenti pone un delicato problema in ordine alla certezza del quadro normativo per operatori e cittadini. La situazione è tanto più delicata in quanto, per ciò che concerne l'ambiente, i valori costituzionalmente tutelati ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 32 meritano una tutela che possa dispiegarsi in piena efficacia sin dalla fase successiva all'approvazione delle leggi di settore. Per quanto concerne le imprese ed in particolare gli operatori dei settori industriale ed edilizio, spesso direttamente interessati alla normativa in ambito ambientale, è nel loro interesse conoscere con chiarezza il quadro della legislazione vigente e degli adempimenti resi obbligatori in forza di legge. In tal modo - come dicevo in premessa - è possibile programmare con rigore e serietà l'attività d'impresa ed assicurare, al contempo, l'attuazione delle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio, cosa che con le proroghe non riusciamo a fare; si sentiranno gabbati. In alcuni casi la proroga è spiegabile e giustificabile, lo è meno quando, come in questo caso, la proroga viene con decreto-legge; decreto che è emanato dal Governo, cioè dalle amministrazioni che dovrebbero applicare le leggi e invece ne dispongono il rinvio (prima si approvano e poi la loro effettiva capacità di essere attive viene rinviata nel tempo). Infine, è censurabile la prassi del rinvio continuo, vale a dire della pratica ormai dilagante di rinviare più volte la stessa legge ad ogni scadere del termine. La reiterazione della proroga comporta, di fatto, la cancellazione della norma (come abbiamo fatto questa mattina con il decreto milleproroghe; ora saranno 1.100, con quelle che stiamo esaminando). Nel caso del decreto-legge in esame, sono numerose le proroghe disposte. In alcuni casi si parla di termini rinviati quando sono già scaduti (fatto ancora più grave), con l'effetto di veder beffati i cittadini e gli imprenditori che si sono fatti cura di osservare le leggi nei tempi e nei modi prescritti. Vi è dunque una situazione complessiva di confusione che non aiuta certamente l'interprete e i cittadini nel comprendere le norme nel loro succedersi coerente. Ma il disegno di legge in esame va oltre le semplici proroghe. In materia di danno ambientale esso modifica l'ordinamento vigente, a fin di bene, dice il relatore, ma in realtà comprimendo i poteri e le competenze di Regioni ed enti locali. L'articolo 2 del decreto-legge, infatti, prevede la possibilità di ricorrere ad una procedura alternativa stragiudiziale per il ristoro dei danni ambientali. La motivazione della norma, stando alla relazione, consisterebbe nel consentire il recupero "in tempi certi" delle aree contaminate e di evitare ogni rischio di diffuso contenzioso. Va segnalato, tuttavia, che la motivazione recata nella relazione illustrativa non pare sostenere adeguatamente le caratteristiche di straordinaria necessità ed urgenza che renderebbero legittimo il ricorso alla decretazione da parte del Governo in materia di danno ambientale, essendo tale ambito già esaustivamente disciplinato dal codice dell'ambiente attualmente in vigore ed essendo da tempo avviate le procedure relative ai siti di interesse nazionale. Vi è semmai la necessità di accelerare, con finanziamenti e autorizzazioni, tali operazioni di bonifica e ripristino, senza incidere sul regime di responsabilità di chi ha contribuito o determinato il sorgere dell'inquinamento. Vi è inoltre la necessità di non sovrapporre le transazioni globali di cui all'articolo 2 con quelle già eventualmente stipulate. Nel merito, si evidenzia come, in base al decreto in esame, il Ministro dell'Ambiente sia autorizzato a stipulare una transazione, definita molto enfaticamente "globale", ma tale possibilità non viene, apparentemente, ancorata a criteri definiti e certi , configurandosi come eventuale e discrezionale. Quindi, Regioni, enti locali interessati, privati e associazioni, possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni, senza avere però - guarda caso - il diritto a ricevere una risposta, come espressamente si premura di specificare la norma con una formulazione che mai abbiamo visto in una legge. In particolare, come ha rilevato la Commissione affari costituzionali in sede di parere sugli emendamenti 2.14 e 2.24, lo Stato non può cancellare danni ambientali che interessano altri enti territoriali, precludendo ad altri ogni ulteriore azione per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria. È comunque essenziale che tali nuove procedure non facciano venir meno, quale effetto di una transazione sulla quale molti soggetti interessati non potranno più incidere, responsabilità e diritti e diritti afferenti a casi assai gravi di danno ambientale. Ciò sarebbe assai grave per vicende di inquinamento e contaminazione più o meno eclatanti, sulle quali è in essere una valutazione della magistratura, non potendosi ritenere accettabile che responsabilità penali siano estinte per il venir meno della controversia sul danno derivante da accordo stragiudiziale. In mancanza di criteri specifici non si comprende, inoltre, quali cautele siano state studiate e poste circa la congruità delle transazioni che verrebbero ad essere stipulate in forza del decreto in oggetto. Per quanto riguarda le proroghe contenute negli articoli successivi, su alcune si può convenire, mentre per altre restano tutte le ragioni di contrarietà già espresse da più parti in sede di esame in Commissione. Valutiamo positivamente, perché necessaria, la proroga per le autorità di bacino, che non sono state ancora sostituite dalle autorità di distretto idrogeografìco, creando dubbi ed incertezze sull'invalidazione degli atti di ordinaria amministrazione per la tutela del territorio. Mi rendo conto che il tempo a mia

Questo non va certamente nel senso da noi auspicato, perché noi siamo per la stabilizzazione di tutti i lavoratori precari. Signor Presidente, il decreto-legge in esame contiene rilevanti e importanti disposizioni di modifica del codice dell'ambiente. esso è disposizione per il finanziamento dei danni subiti dal Paese in occasione delle ultime calamità naturali. Gran parte del territorio nazionale è a rischio idrogeologico e sono evidenti i disastri provocati ogni anno dalle alluvioni che mettono in ginocchio le valli del Nord, le aree più produttive del Paese, e creano disastri ciclici, allagamenti, inondazioni, frane e dissesti di varia natura su tutto il territorio nazionale. L'articolo 8 del decreto autorizza, infatti, la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eventi alluvionali che negli ultimi mesi hanno interessato gran parte delle Regioni e del territorio nazionale, causando danni diffusi e, purtroppo, il decesso di otto persone. Si tratta degli ultimi danni causati dagli eventi alluvionali che appartengono a una serie di fenomeni che si ripetono, purtroppo, ogni anno. Ma l'intervento di emergenza non deve diventare la prassi, com'è avvenuto negli ultimi tempi. Occorre una progressiva maturazione di diffuse sensibilità che portino al generarsi di nuovi equilibri tra azioni sul territorio, stili di vita, strategie efficaci di sviluppo sostenibile ed utilizzazione razionale delle risorse naturali. La scarsità di risorse finanziarie, da una parte, l'attuazione del Patto di stabilità, dall'altra, che impedisce agli enti locali di escludere dal Patto stesso le risorse finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico (fatto salvo solo il caso dell'avvenuta dichiarazione di calamità naturale), rendono assai esigue le risorse ordinarie destinate all'azione della prevenzione del rischio idrogeologico. A ciò si aggiunge la cattiva gestione dei bacini idrografici e la sovrapposizione di competenza tra varie autorità, centrali e locali, che mettono in pericolo il corretto ed efficace svolgimento della salvaguardia del territorio. le autorità di bacino, così come concepite, oggi non funzionano. La garanzia della permanenza dei poteri fino alla riforma, come proposto dal presente decreto-legge, è un atto dovuto per evitare mali peggiori. Come è un atto dovuto anche l'emendamento del relatore che agevola il coordinamento per l'adozione dei piani di gestione, come previsto dalle direttive comunitarie. Ma la vera riforma della materia della difesa del suolo deve prevedere un riordino radicale delle competenze dei bacini idrografici, prima di tutti di quello del fiume Po, che attraversa il territorio di ben quattro Regioni. Infatti, per quanto riguarda il Po, in attesa della istituzione effettiva dell'autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico padano, le competenze relative alla pianificazione territoriale, alla programmazione degli interventi e alla definizione della vincolistica sono esercitate dall'autorità di bacino del Po, istituita ai sensi della legge n. 183 del 1989. Nello stesso bacino padano, per l'esercizio delle funzioni trasferite alle Regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, è stata istituita l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), tra le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, che opera soprattutto in materia di progettazione ed attuazione di interventi idraulici fluviali, di polizia idraulica e del servizio di piena, nonché di navigazione interna. L'autorità di bacino e l'AIPO fanno - come si è visto -riferimento a due «livelli» di norme che appaiono disgiunte e che non necessariamente sono agevolmente integrabili. Situazioni analoghe di accavallamento di competenze si verificano su tutti i bacini idrografici nazionali. Il nostro Gruppo ha presentato un emendamento con l'obiettivo di ottimizzare l'azione complessiva della pubblica amministrazione, evitando sovrapposizioni ed azioni non coordinate. La nostra proposta prevede che le Agenzie regionali (e l'AIPO, per quanto riguarda il fiume Po) diventino parte integrante della struttura di distretto, pur rimanendo controllate e gestite dalle Regioni. L'articolazione individuata porta alla creazione di un unico soggetto competente per ciascun bacino idrografico, in materia di difesa del suolo, dalla programmazione all'attuazione e gestione degli degli interventi, con incremento di efficienza, di efficacia e di economicità nelle varie azioni da porre in atto. Purtroppo l'emendamento non è stato approvato dalla Commissione, anche per il parere contrario della 5a Commissione, che ha riscontrato la creazione di maggiori oneri dovuti all'articolazione delle competenze tra sezione centrale e sezioni periferiche. Il nostro Gruppo presenterà in altre occasioni la proposta emendativa che individua una soluzione radicale al problema delle sovrapposizioni delle competenze nell'ambito dello stesso bacino Il Gruppo esprime comunque soddisfazione per l'approvazione in Commissione di un altro nostro emendamento che destina ad interventi di difesa del suolo i finanziamenti (pari al 10 per cento delle risorse complessive) che attualmente vengono destinati alle attività di studi e progettazioni per la predisposizione dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio. tutte già approvato i PAI, non si ritiene utile destinare ancora risorse per progetti e studi, volendo piuttosto favorire la realizzazione di opere di difesa del suolo. Ciò anche in considerazione delle carenze emergenti ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico. Di grandissimo rilievo per l'ambiente, per il mondo imprenditoriale e per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio è l'articolo 2 del decreto-legge, che interviene nella materia delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), attraverso una nuova disciplina sul «danno ambientale». Il testo intende risolvere l'inconcludente contenzioso pendente sul risarcimento del danno ambientale con un unico contratto transattivo. Si tratta di un obiettivo condivisibile per dare certezza agli imprenditori e permettere il riutilizzo dei siti contaminati. Infatti, attualmente, numerosi progetti di investimento che riguardano siti di interesse nazionale sono bloccati sia per il contenzioso pendente, sia per la mancanza delle autorizzazioni, sia a causa delle prescrizioni per le procedure di bonifica impartite dal Ministero dell'ambiente, che spesso chiedono modifiche di progetti di bonifica già approvati o già in parte realizzati. La situazione si presenta alquanto critica per le imprese che vedono bloccati cospicui investimenti industriali, importantissimi per il rilancio industriale delle aree. Occorrono interventi urgenti indirizzati: a portare a termine gli interventi di bonifica, a costi sostenibili e con criteri procedurali certi; a sbloccare i progetti di investimento, rilanciando le aree industriali; a porre a carico delle aziende responsabili dell'inquinamento i costi della riparazione del danno ambientale. Vorrei esprimere la soddisfazione del nostro Gruppo su una disposizione fondamentale approvata dalla Commissione 13a su un emendamento della Lega Nord, riformulato dal relatore, che fa finalmente chiarezza sull'applicazione delle norme che regolano le immissioni di rumore in una proprietà privata. Il caso dell'autodromo di Monza è la dimostrazione più eclatante della situazione contraddittoria che si è venuta a creare fino ad oggi, a causa dell'applicazione indiscriminata dell'articolo 844 del codice civile, che dimostra come un gruppo minoritario di appena otto persone, su circa 1.700 residenti nelle vicinanze (che, intervistati, hanno escluso qualsiasi fastidio), sia riuscito a mettere a rischio l'attività dell'autodromo, basandosi su principi di natura esclusivamente soggettiva e in contrasto con le norme e i regolamenti che disciplinano l'inquinamento acustico legge n. 447 del 1995 e i successivi decreti attuativi), che impongono norme severe ma eque per tutelare i cittadini dal rumore, anche tenendo conto delle zone territoriali di insediamento delle sorgenti sonore. È nota a tutti la storia dell'autodromo, costruito nel 1922, ben prima che i cittadini ricorrenti si insediassero nelle zone limitrofe allo stesso autodromo. Ed è sotto gli occhi di tutti l'importanza mondiale di tale circuito italiano, sia per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, sia per le diverse manifestazioni sportive e le prove di autovetture e moto. Con l'approvazione del nostro emendamento, il mero principio giurisprudenziale dell'identificazione del concetto di «normale tollerabilità» con la soglia dei 3 decibel (di provenienza «pseudoscientifica»), che non tiene conto della zonizzazione acustica comunale, delle caratteristiche della zona, delle attività prevalenti nella zona e del valore del «rumore di fondo», non può prevalere sulle leggi dello Stato che, puntualmente, negli ultimi anni hanno definito la disciplina

stanzia 19 milioni di euro per i danni del terremoto che ha colpito le Province di Parma e Reggio Emilia il 23 dicembre scorso. Tali risorse si aggiungono ai 15 milioni di euro promessi dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Protezione civile e sono destinati a far fronte ai primi interventi emergenziali del post-terremoto. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il decreto al nostro esame prevede, tra le altre, disposizioni riguardanti la Protezione civile, l'autorizzazione di spesa per 100 milioni di euro da assegnare al Dipartimento della Presidenza del Consiglio per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito nei mesi scorsi il territorio nazionale, nonché l'obbligo della rendicontazione previsto per i commissari delegati titolari di contabilità speciali entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e al termine della gestione dell'incarico (rendicontazione delle entrate, delle spese, delle tipologie dei soggetti beneficiari). Bene la trasparenza. Manca totalmente, azzerato dalla legge finanziaria per il 2009, il fondo regionale di Protezione civile, non più rifinanziato per l'anno 2009 e seguenti, una decisione gravissima che toglie alle Regioni qualsiasi possibilità di intervento urgente conseguente alle calamità naturali. È come dire ai cittadini: «Vi lasciamo soli». Nel corso dei lavori in Commissione il dibattito si è intrecciato con audizioni del sottosegretario Bertolaso, sempre più condizionato, come capo della Protezione civile, dalle scelte del Governo.

Entrambe hanno messo in luce il cuore del problema: la Protezione civile è una struttura fondamentale per il Paese e sta a cuore a tutti gli italiani. Grande deve essere l'investimento per renderla sempre più adeguata; ma, nello stesso tempo, grande deve essere lo sforzo del Governo e del Parlamento per affrontare i problemi strutturali dell'assetto idrogeologico del Paese, investendo sulla prevenzione. Non basta il dottor Bertolaso, puntuale ed efficace quando avvengono le calamità; occorre un'altra politica, con ben altri investimenti.

Il sisma è stato serio: magnitudo 5,1, profondità 27 chilometri. Ha coinvolto molti comuni; più di 150 famiglie evacuate, edifici privati inagibili, scuole, municipi, chiese, castelli, di Torrechiara in Provincia di Parma e di Bianello in Provincia di Reggio Emilia, lesionati seriamente. L'intervento del sistema di Protezione civile nazionale, regionale e locale è stato esemplare per tempestività, intelligenza, organizzazione.

in esame, grazie ad emendamenti dei parlamentari accolti dal Governo, si aggiungono ulteriori 19 milioni di euro. Bene. Noi del Partito Democratico ne avevamo chiesti e ne chiediamo un po' di più, almeno una trentina. Il problema è proprio questo: si stima un danno complessivo di almeno 150 milioni di euro; questa è la sproporzione. Si deve intervenire subito per recuperare gli edifici danneggiati. Le chiese, soprattutto, che sono circa 200, senza un tempestivo intervento rischiano ulteriori danni, quale il crollo, ed hanno quindi bisogno di un tempestivo intervento pubblico. Lo sottolineo perché esse appartengono al patrimonio civile e non soltanto religioso delle nostre comunità.

con risorse e agevolazioni, alle famiglie colpite. Si devono agevolare, anche in rapporto al Patto di stabilità, i Comuni colpiti, i cui sindaci sono stati dal primo momento impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza. Oggi è tempo di dare maggiori sicurezze ed è tempo di aprire una fase nuova. Lo abbiamo detto in Commissione e lo ha ricordato il relatore. Bisogna investire sulla prevenzione, su un piano pluriennale di prevenzione, in un progetto a lungo termine, perché in Italia i terremoti sono ricorrenti e perché nella zona di Parma e Reggio Emilia lo sono ancora di più. Si deve anche sapere che se in questo evento sismico non vi sono state vittime, a differenza di quanto sarebbe potuto accadere in altre aree del Paese, lo si deve al sistema abitativo dell'Emilia Romagna, che da tempo ha provveduto ad adottare i criteri di prevenzione antisismica. Occorre continuare a recuperare e a consolidare per evitare problemi peggiori. Per questo riteniamo che i fondi fino ad ora stanziati, ancorché utili, siano insufficienti. Ed è per questo che anche in Aula indichiamo, con la presentazione di un emendamento e di un ordine del giorno, la necessità che il Governo assuma l'impegno di deliberare un investimento maggiore, al fine di dare continuità agli investimenti di prevenzione, di consolidamento e di messa in sicurezza. Non possiamo rincorrere i problemi: dobbiamo prevenirli e risolverli meglio. Il Governo, il Parlamento, le Regioni, le autonomie locali sono un sistema, l'unico sistema che può governare il territorio e affrontare finalmente un piano organico per mettere in sicurezza tutto l'assetto idrogeologico del Paese. La situazione è seria, sappiamo che siamo in presenza di zone a crescente rischio sismico, di nuove condizioni meteorologiche che alternano siccità, forte innevamento e piogge copiose, mettendo a rischio il nostro territorio, l'Appennino e la pianura. Pensiamo seriamente ad affrontare "il" problema: non basta una manciata di milioni di euro soltanto nell'emergenza, dobbiamo sentire la responsabilità di rilanciare il Paese anche provvedendo in tema di sicurezza ambientale e territoriale. La vita dei cittadini dipende anche da questo. Ed è su questo terreno, che non è per nulla secondario rispetto ad un nuovo sviluppo dell'Italia e alla sua crescita, che mi auguro che la maggioranza e l'opposizione possano insieme confrontarsi per scelte positive nell'interesse del Paese, oggi nell'emergenza, ma guardando più in là.

provvedimento, il relatore, che è anche il presidente della Commissione ambiente, il senatore D'Alì, e tutti i membri della 13a Commissione, perché intorno a questo disegno di legge si è sviluppata un'ampia discussione. avviso, testimonia quanto lavoro ci sia da fare in tema di legislazione ambientale, in modo assolutamente trasversale, rispetto alle tante situazioni situazioni che richiedono di trovare un punto di equilibrio tra le attività dei cittadini, l'attività delle imprese e i risvolti di carattere ambientale. Ciò testimonia inoltre come sia davvero maturata, nella nostra società, nella nostra comunità, la sensibilità rispetto ai temi ambientali. Con grande soddisfazione,

una soluzione a temi che spesso, da tempo, non trovano risposte.

non è così facile costruire un ragionamento politico complessivo su una norma che, come già è stato detto in quest'Aula, è la sommatoria di tante esigenze e criticità. un ragionamento complessivo che non si può fare, ma che può essere in qualche modo sintetizzato dal bisogno diffuso di semplificazione normativa sulle tematiche ambientali, Certo, abbiamo la consapevolezza che con questo provvedimento non stiamo dando una risposta a tutte le questioni. Molte delle questioni affrontate in Commissione, man mano che venivano approfondite, aprivano scenari complessi e di non semplice soluzione. Credo che ciò debba spronarci a lavorare in Commissione in maniera approfondita su molte delle tematiche che sono emerse come particolarmente sentite dai settori produttivi del Paese, ad esempio. Proprio nel momento in cui c'è una grande richiesta di sostegno all'economia, è evidente che questo sostegno lo si può costruire non solo con interventi di carattere finanziario, ma lo si può e lo si deve costruire anche con interventi di carattere semplificatorio dal punto di vista normativo. E uno dei risvolti che nelle norme purtroppo così diffuse e oggetto di proliferazione nel nostro Paese crea problemi nei settori produttivi è proprio l'aspetto ambientale. Da questo punto di vista, ad esempio, il tentativo evidenziato nel provvedimento di porre mano alle questioni legate al danno ambientale e ai contratti di transazione rappresenta un tentativo di consentire interventi di sviluppo in territori e in aree industriali che non siano state toccate dal danno ambientale. Esso consente, alle parti interessate alla composizione del danno ambientale che si è creato di arrivare con tempi più rapidi ad una definizione, con soddisfazione del ristoro ambientale del territorio dei danni subiti e con l'avvio di incisivi interventi di bonifica. Questo emerge nei vari emendamenti (ad esempio, nell'emendamento 2.390) nei quali si è cercato di definire al meglio queste procedure, consentendo anche, a quegli imprenditori che sono proprietari di aree che non sono state state toccate da inquinamento ambientale ma sono perimetrate all'interno dell'area di interesse nazionale, di poter attuare investimenti coerentemente con le previsioni urbanistiche del Comune nel quale è localizzata quest'area. Ho sentito criticare la questione delle proroghe. Certo, è naturale che in quest'Aula si evidenzi la criticità del metodo delle proroghe, però credo che dobbiamo domandarci perché nel nostro Paese c'è così spesso il ricorso alle proroghe. Probabilmente c'è anche una legislazione velleitaria: se il Paese reale non riesce a star dietro alla legislazione, non è perché è pigro; forse spesso noi legiferiamo in maniera eccessiva rispetto alle reali capacità; forse pensiamo più ad un approccio ideologico e alla speranza di realizzare in tempi rapidi delle trasformazioni anche sociali del nostro Paese che a quello che in realtà il sistema può realizzare. Questo aspetto appare particolarmente evidente, ad esempio, nell'argomento trattato nell'emendamento 5.200 del Governo, nel quale si pone mano a una proroga rispetto agli obblighi assunti in sede comunitaria di divieto di smaltimento in discarica di determinate tipologie di rifiuti. Questo tocca

problemi che verrebbero fuori e che emergono dall'applicazione di questa norma a cui siamo obbligati per impegni assunti in sede europea e per evitare l'apertura di contenziosi

tutti i componenti in metallo recuperabili, ad esempio in impianti di termovalorizzazione perché, come ben sapete colleghi, c'è una pregiudiziale fortissima, in tutte le comunità locali, rispetto alla localizzazione di impianti tecnologici di questo tipo. Anche i Comuni, nelle forme consortili nelle quali si organizzano per gestire le frazioni di raccolta differenziata o meno, trovano difficoltà a realizzare impianti di termovalorizzazione. È allora evidente che non facciamo proroghe per una brutta

la tariffa rifiuti urbani. È già intervenuta sul tema la collega Mazzuconi evidenziando come sia più corretto un approccio a tariffa rispetto ad un approccio a tassa, che ancora esiste in un numero significativo di Comuni del nostro Paese. Con questo emendamento ho evidenziato quanto sarebbe ancora più equo che la suddivisione dei costi tra i cittadini avvenisse non sulla metratura, o comunque su un parametro che è anche quello della metratura, ma sul parametro cosiddetto *pro capite* perché, come ben sanno i colleghi, la produzione di rifiuti non è effettuata dai metri quadri dell'abitazione ma dalle singole persone: siamo a circa a 500 chili di rifiuti l'anno *pro capite* prodotti.

Sono diversi gli argomenti che in questo disegno di legge abbiamo trattato. Non è certo un provvedimento esaustivo della grande domanda di semplificazione il Paese, dai singoli cittadini alle categorie produttive, ci pone in termini di politica ambientale. Sono pochi mesi che il nostro Governo è al lavoro; il Ministro sta ben operando in questa direzione.

piena consapevolezza dell'importanza dei temi ambientali, ma altrettanta piena consapevolezza che questi non possono più essere affrontati in modo ideologico, come lo è stato per anni da parte della sinistra ambientalista, provocando molti danni al nostro Paese ed alle nostre comunità.

Presidente, aggiungerò solo qualche parola. Tra l'altro, la relazione del Presidente della Commissione, in questo caso anche relatore del provvedimento, è stata ampia, esaustiva, convincente e puntuale. Da parte dell'opposizione sono arrivate anche una serie di critiche, come è logico, legittimo e doveroso. Sotto altro profilo, devo anche dire che la Commissione su questo provvedimento ha lavorato in modo egregio. Tra l'altro, in Commissione una serie di emendamenti che giungevano tanto dall'una quanto dall'altra parte

perché comunque riguarda questioni ambientali ed urgenti ed in alcuni casi mi pare indubitabile la necessità di intervenire Mi riferisco soprattutto alle norme dell'articolo 1, relative alla sopravvivenza delle autorità di bacino.

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 1.5 parere non ostativo, ritenendo necessario, al capoverso 6-*quinquies*, prevedere un'intesa con le Regioni interessate all'interno della procedura di trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie delle Agenzie regionali e interregionali alla Conferenza interregionale di indirizzo; - sugli emendamenti 2.8, 2,9, 2.10, 2.11 e 2.36 parere favorevole, poiché opportunamente prevedono l'intesa, in sede di Conferenza unificata, sia nella predisposizione dello schema di contratto di cui all'articolo 2, comma 1, sia per la riassegnazione dei proventi derivanti dalle transazioni di cui al comma 7 del medesimo articolo 2; sull'emendamento 2.400 parere non ostativo, ritenendo opportuno prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata nella fase di adozione del decreto ministeriale che definisce tipologie, quantità, qualità e modalità di raccolta dei rifiuti; sull'emendamento 5.200a parere non ostativo, invitando a valutare se, all'ultimo periodo del capoverso 1-*ter*, non si configuri una possibile lesione dell'autonomia tributaria degli enti locali; sull'emendamento 7.0.7 parere non ostativo, invitando a verificare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione delle modalità di diffusione degli aspetti contenutistici

Nonostante ci sia un autorevole parere che mi è venuto a riferire il senatore Ferrara, io sono però legato agli orientamenti del Presidente del Senato. Quindi, o c'è silenzio, o stiamo qui fino a quando non ci sarà un silenzio che consenta alla senatrice Thaler Ausserhofer di poter leggere tranquillamente questi pareri. sull'emendamento 8.0.12 parere non ostativo, rilevando l'opportunità dì sopprimere il comma 7 che, oltre ad essere lesivo delle competenze costituzionalmente

in riferimento al giudizio di compatibilità ambientale emesso, per competenza, dalle Regioni e dalle Province; - sugli emendamenti 8.0.203 e 8.0.204 parere non ostativo rilevando l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nella redazione del documento tecnico previsto per i dragaggi in aree portuali; - parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

Stato - del maggior gettito IVA». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi ai disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 2.23, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.37, 2.38, 2.0.1, 5.300/3 (limitatamente alla lettera 6.3 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.4 (limitatamente al capoverso 1-*bis*, lettera a), 6.5 (limitatamente al capoverso l-*bis* lettera 7.0.3, 7.0.4, 8.0.5, 8.0.17, 2.0.200, 6.200, 6.0.6, 6.0.7, 8.0.200 e 8.0.21. Esprime parare di semplice contrarietà sulle proposte 8.1, 8.2, 8.500, 8.203 e Esprime parere non ostativo sulla restanti proposte, ad eccezione della proposta 8.0.203, sulla quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo a che, dopo il comma 1, sia inserito il comma 1*-bis* del seguente tenore: ai membri della Commissione di cui al comma 1 non sono riconosciuti compensi o indennità».

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri nell'articolo 1, Tenuto conto poi dei chiarimenti forniti dal Governo sull'articolo 5, in base ai quali la proroga dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) alla tariffa integrata ambientale (TIA) non determina effetti finanziari negativi sul gettito dei Comuni a legislazione vigente, in quanto i Comuni non hanno ancora previsto nei loro bilanci il passaggio al nuovo regime tariffario. La Commissione richiama, tuttavia, l'esigenza di osservare in modo più puntuale il rispetto del criterio della legislazione vigente per la costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Tale criterio implica che il tendenziale rappresenti gli andamenti futuri di finanza pubblica, che si realizzerebbero qualora nulla risulti modificato legislativamente rispetto al momento in cui si effettua la previsione. Il rispetto di tale criterio, in vista di eventuali future proroghe, richiederebbe la previsione, nei bilanci degli enti citati, del passaggio al nuovo regime della TIA a partire dal bilancio per l'anno 2010 in base alla nuove disposizioni di cui all'articolo 5, nonché - nel bilancio dello Stato - del maggior gettito IVA». «La 1a Commissione permanente, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 2.23,

avverto che sono inammissibili per estraneità alla materia trattata dal disegno di legge in esame gli emendamenti che prevedano l'istituzione di nuovi organismi ministeriali rechino modifiche alla disciplina relativa al conferimento di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego. Dichiaro pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) del relatore, 6.0.70 e 8.0.50 della Commissione.

che, in parte, risolveranno il problema evidenziato dai presentatori dell'ordine del giorno in questione, ritengo che il Governo lo possa accogliere come raccomandazione, inserendo la parola «ulteriori» prima della ripeto, in Commissione abbiamo già approvato un emendamento per intervenire con maggior forza sul problema dei

Presidente, gli emendamenti da me presentati sono tesi ad affrontare un problema cui tutti dovremmo essere sensibili che è quello dei tempi necessari per l'approvazione delle opere pubbliche e per l'ottenimento delle autorizzazioni per le per le esecuzioni di infrastrutture. In un momento di crisi come l'attuale, la lotta alla burocrazia è un impegno su cui dovremmo sentirci coinvolti in quanto i ritardi nell'acquisizione di permessi e autorizzazioni impediscono l'avvio di opere che potrebbero dare fiato all'economia. In campagna elettorale tutti gli schieramenti hanno posto alla base dei propri programmi questo impegno. Giova ricordare a tal fine lo slogan "Apriamo un'impresa in un giorno". Per esemplificare i concetti sopra esposti, basta ricordare che tutte le opere, in generale, comportano tempi biblici per l'approvazione e tempi ragionevoli per l'esecuzione. È di questi giorni l'inaugurazione del passante di Mestre, opera che si è sbloccata con la legge Obiettivo, per la cui approvazione sono stati necessari ben sette anni mentre per l'esecuzione soltanto quattro. Gli emendamenti dall'1.200 all'1.212 modificano gli articoli 20, 21, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tendono, nell'insieme, a dimezzare i tempi delle procedure per l'approvazione dei progetti sottoposti a VIA. Gli articoli modificati riguardano la verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, studio di impatto ambientale, la presentazione dell'istanza, la consultazione, la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione e, infine, la decisione. L'emendamento 1.213, a mia firma, prevede una modifica all'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, estendendo la facoltà di non aderire al gestore unico del servizio idrico, previsto dalla cosiddetta legge Galli, anche per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; la norma vigente prevede che tale facoltà sia consentita ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. L'applicazione di questa norma ha dato buoni risultati e ha consentito, soprattutto ai Comuni montani con buona dotazione di acqua potabile, di gestire autonomamente il servizio idrico, con ricadute positive sui cittadini relativamente alle tariffe. È noto a tutti che l'applicazione della legge Galli ha creato grandi problematiche, soprattutto nei centri montani dove l'acqua è considerata quasi un bene naturale; quindi i cittadini di montagna con grande difficoltà accettano di essere equiparati con tariffa d'ambito a quelli residenti nei centri urbani con popolazione rilevante. L'applicazione, quindi, della norma vigente è stata molto apprezzata da quei Comuni che, pur aderendo all'ambito,

Grazie,

presentati dal senatore Zanetta hanno sicuramente un lodevole intendimento, quello di ridurre quanto più possibile alcuni tempi autorizzativi

per l'emendamento 1.213, in quanto la materia ricade in un più complesso riordino di tutta la gestione degli ambiti idrici, che in questo caso viene affrontata per alcune emergenze, ma dal punto di vista strutturale sarà affrontata sicuramente in un prossimo disegno di legge

la Commissione VIA, negli ultimi mesi, ha smaltito molto lavoro arretrato, così dimostrando che, a prescindere dall'attuale regime e dall'attuale tempistica, si può anche lavorare.

sul codice ambientale, nel momento in cui è stato affermato dal Ministro di volere intervenire in sede emendativa con un provvedimento organico, il Governo è tendenzialmente sfavorevole ad intervenire con emendamenti con emendamenti che, in particolare, tocchino l'uno o l'altro campo ma senza organicità. Questo è il motivo per il quale, su questi e su altri emendamenti (che abbiano magari le loro nobili ragioni), il Governo è sempre intenzionato a dire no, un no che può diventare un invito al ritiro e alla presentazione di ordini del giorno, nel momento in cui condivida le finalità degli stessi. Questo è ciò che mi interessava

Signor Sottosegretario, non capisco come si possa procedere all'approvazione di tali norme, in un momento in cui in molte aree del Paese è necessario procedere ad una bonifica e in altrettante altre la bonifica non è stata fatta a regola d'arte. Vorrei far notare ai colleghi della maggioranza come con questo articolo si prevede l'abbandono del contenzioso e dunque la rinuncia al diritto di far valere le proprie legittime pretese da parte di enti locali pubblici territoriali, anche se gli stessi non sono contemplati come parti nella stipula del contratto di transazione, con ciò venendo meno all'inviolabile diritto alla difesa di cui all'articolo 24, comma 1, della nostra Costituzione. Si potrebbe con ciò sottovalutare sia il danno ambientale, sia la salvaguardia del diritto alla salute da parte dei cittadini. Con questo articolo si rischia di chiudere qualsiasi contenzioso penale e civile sul danno ambientale attraverso una una risoluzione stragiudiziale, cioè un contratto che impedisce ai cittadini e alle istituzioni lese dal danno ambientale di rivalersi su chi ha inquinato. Credo che tutti noi dobbiamo stare attenti a non fare una sanatoria e un regalo a chi ha inquinato. Vorrei che il Governo dedicasse una particolare attenzione

L'obiettivo degli emendamenti che ho presentato è quello di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'articolo 2, che - così com'è scritto - ha un'estensione eccessivamente ampia, e soprattutto coinvolgere pienamente nella procedura che viene prevista le Regioni e gli enti locali che - come ho detto già in discussione generale e come ha ricordato la collega Bianchi - rischiano di

2.130 risponde all'esigenza manifestata in Commissione, dopo un lungo dibattito, di dare pubblicità alle osservazioni fatte pervenire da chiunque sia interessato a questo schema di contratto, prevedendo che tali osservazioni siano rese note ai partecipanti alla Conferenza che deve decidere sull'approvazione o reiezione dello stesso schema di contratto.

«A tal fine, alla stipula della transazione partecipano altresì, senza che ad essi possano essere imputati oneri connessi alla bonifica, al ripristino e al risanamento del danno ambientale, i proprietari dei terreni ricompresi nel sito che dovessero risultare non inquinati e non responsabili dell'inquinamento delle falde».

norma porzioni di terreno che nell'ambito di un sito inquinato non siano inquinate e quindi non debbano intervenire nelle operazioni di bonifica del sito.

Si rende anche necessario, consequenzialmente, che tale previsione sia estesa a terreni che di per sé non hanno mai avuto autonomamente alcuna traccia di bonifica o non abbiano mai partecipato alla bonifica e che comunque siano ricompresi in una perimetrazione del sito inquinato. Questi terreni resterebbero in un limbo, non sapendo se, una volta

proventi derivanti da somme di risarcimento (quindi non solo da somme necessarie all'attività materiale di bonifica, ma relative

un vantaggio nell'esazione dei crediti attraverso ruoli, quasi si trattasse di imposte dirette a favore dello Stato anziché, come si tratta, di contributi a favore di organismi la cui stessa natura è stata inquadrata e definita in modo diverso.

Ho provato poco fa ad indicare la motivazione di quella modifica. I siti inquinati molto spesso sono individuati con un ampio raggio e possono ricomprendere anche terreni che non sono inquinati all'interno di quei siti

La partecipazione di tutti i terreni e, quindi, dei proprietari dei terreni inseriti in un sito inquinato ritengo risponda anche ad un interesse generale:

Questa formulazione, quindi, lascia un'incertezza molto ampia e consente anche che proprietari di terreni accedano a contratti transattivi per condividerne i benefici quando non ne avrebbero titolo.

2.12 potrebbe essere accolto solo nella seconda parte e modificando le parole «impresa interessata» con le altre «imprese interessate».

e 2.22 c'è un invito al ritiro.

ha presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2. Vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su cosa stiamo votando. Noi stiamo votando una procedura transattiva che chiude ogni possibile contenzioso per le aree e per i siti di interesse nazionale per quanto concerne gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza. Il Partito Democratico non è contrario a trovare una modalità transattiva per chiudere una serie di questioni che sono aperte, ma questo articolo è frettoloso

abbiamo soggetti privati che hanno cambiato ragione sociale e abbiamo soggetti privati che sono falliti. Il non prevedere in nessun modo l'articolazione che riguarda tutta questa materia è sbagliato e rischia di portarci a una sorta di condono tombale con questi schemi che vengono prodotti centralisticamente. Già in Commissione ho avuto modo di dire al relatore ed al rappresentante del Governo che forse una una normativa più cauta, più articolata e anche più precisa rispetto alle varie situazioni ci avrebbe trovato d'accordo. Così non è stato.

e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo. Ma se queste risorse di bilancio non ci sono, chi ne informa,

successivamente si dice che "i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta". E solo a seguito di insistenze notevoli svoltesi in Commissione, si è trovata una formula che prevede le osservazioni verranno fatte circolare, ma non si capisce chi tenga conto delle osservazioni fatte pervenire da soggetti interessati. Non parlo solo dei privati interessati, ma anche di tutti i soggetti pubblici. Quindi, con molta franchezza, il Partito Democratico non può votare questo articolo che verte - torno a ripetere - su un problema vero e reale, ma che in maniera troppo frettolosa di fatto rischia di fare più danni di quanti non ne voglia risolvere. Meglio sarebbe stato sui casi già pronti per una transazione chiamare questi casi per nome e cognome e dire che per questi si avviava quella procedura. Dire che questa procedura è generalizzata è un errore, creerà problemi, e noi ci ritroveremo sicuramente in questa Aula a ridiscutere di tali questioni, ma soprattutto della questione che non ci può essere un condono tombale. Come facciamo a dire ci sarà l'abbandono di ogni contenzioso pendente e che la stipula del contratto preclude ogni ulteriore azione per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, senza dire che il danno ambientale è noto nel momento in cui viene stipulata Non è possibile. Molti di questi siti sono delle vere e proprie discariche industriali e noi non sappiamo quando gli effetti disastrosi continueranno a far sentire le loro conseguenze o quando questi effetti disastrosi cesseranno. Quindi, dico che siamo disponibili a discutere di transazione, ma su di essa bisogna discutere con calma, capire i casi e verificare tutte le ipotesi possibili perché a gravi danni ambientali - ricordo che sono siti di interesse nazionale - non si aggiungano ulteriori e più gravi danni per il territorio e per l'ambiente.

pone non solo a noi, ma al Paese, soprattutto in una materia così delicata come il rispetto dell'ambiente e la bonifica di aree altamente degradate.

Il tema dei siti di interesse nazionale è particolarmente complesso e delicato. La voce "danno ambientale" è particolarmente sfumata in questa lettura che possiamo fare.

2.270, laddove prevede che "sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati". Nel momento in cui si usa l'aggettivo "transattivo" si fa chiaramente riferimento al 1969 ed alle reciproche concessioni, quindi si esclude

Presidente, credo sia necessario riportare la discussione sul contenuto dell'articolo 2, che poi è il cuore di questo provvedimento, alla sua portata, alle sue buone ragioni ed alle motivazioni fortemente utili dal punto di vista ambientale che hanno prodotto tale norma. Molti colleghi che sono intervenuti hanno omesso di ricordare che l'articolo 2 si applica negli ambiti di approvazione dei progetti di bonifica. Vi è quindi un soggetto che si è reso disponibile ad effettuare una bonifica, secondo un progetto che viene approvato da una Conferenza dei servizi, quasi sempre coordinata dal Ministero dell'ambiente. Questo soggetto, che assume l'obbligo della bonifica e che lo pone in essere, o è messo in condizione di sapere che realizzando la bonifica stessa, come il progetto approvato dalla pubblica autorità gli impone, non avrà altre pendenze, oppure attende, come purtroppo sta accadendo dopo una nefasta azione del precedente ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio nei confronti di tutti i soggetti presunti responsabili di attività di inquinamento, il giudizio di secondo grado, nel quale verrà condannato ad effettuare la bonifica che liberamente si assume come obbligo nell'ambito di una procedura concertativa.

da tutte le altre nelle quali non vi è un soggetto che si assume questo obbligo (che è giusto perseguire, e che si continuerà a perseguire nell'ambito dell'articolo dell'articolo 2), oppure affidiamo ai tempi della giustizia ordinaria la certificazione e la verifica dell'obbligo di bonifica da parte di soggetti che oggi si rendono disponibili ad effettuarla. È per questo che sosteniamo tale provvedimento con il quale ripartiranno le bonifiche nel nostro Paese. Pensate a tutte le bonifiche presentate dall'ENI e dalle società pubbliche, che assumono nei loro bilanci gli obblighi di ripristino ambientale, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità giuridica, ma non di una responsabilità morale.

quando un soggetto, quello ritenuto responsabile, assume integralmente l'obbligo della bonifica. A tale soggetto credo che dobbiamo prestare attenzione. Al soggetto che farà la bonifica, secondo il progetto approvato dalla pubblica autorità, ossia dal Ministero dell'ambiente, dobbiamo anche offrire la possibilità e la certezza che, oltre al ripristino ambientale che gli viene richiesto, non sarà soggetto ad ulteriori procedimenti ed azioni di tipo risarcitorio. Con l'avvio e la denuncia di danno ambientale, indiscriminatamente per tutti i siti di interesse nazionale, attivata dal precedente Governo, noi abbiamo fermato le bonifiche in questo Paese, anche quelle che - lo ripeto - avevano un soggetto che si era assunto Per questo motivo, l'articolo 2 è utile all'ambiente; è utile all'economia perché libera grandi risorse nei confronti di settori che investiranno, faranno ricerca e recupereranno aree; è utile a recuperare delle aree all'uso produttivo e quindi poterle destinare e programmare; è utile a superare una situazione di incertezza e di stallo che caratterizza la quasi totalità dei siti di interesse nazionale e la gran parte dei siti accertati come inquinati, indipendentemente vi sia qualcuno che tenta di fuggire dalle proprie responsabilità o se invece c'è qualcuno che si assume le proprie responsabilità, mette mano al portafoglio e rimedia ai danni provocati.

**Il Senato non approva.**

inquina paga», e dopo le parole: «schema di contratto, che viene», inserire le seguenti: «concordato con l'impresa interessata

che chi inquina paga». Allora, da questo si vede quali sono le intenzioni reali che stanno dietro queste modalità transattive. Io non aggiungo altro.

**Il Senato non approva.**

Governo

e poi due emendamenti modificativi che sono stati accolti in una riformulazione del relatore che la Commissione ha votato all'unanimità: si tratta dell'emendamento 5.41.

ove il Ministro non preveda entro il 30 giugno di quest'anno a fare il regolamento applicativo previsto dal decreto n. 152 del 2006, i Comuni che siano pronti e che lo desiderino possono passare al

Presidente, io illustro soltanto l'emendamento 5.300/101, che è un subemendamento all'emendamento 5.300, presentato dalla Commissione. Il tema è molto delicato e meriterebbe un po' di attenzione da parte del Governo e della maggioranza. Sostanzialmente, con questo emendamento presentato dalla Commissione si concede una proroga indifferenziata e automatica a tutte le discariche di rifiuti inerti o urbani non pericolosi. Formalmente, non si tratta di una proroga automatica perché si dice che le Regioni e i Comuni devono presentare una richiesta entro il 15 marzo del 2009 e che a questa richiesta deve essere data risposta entro il 31 marzo 2009. Ora, è evidente a tutti che 15 giorni di intervallo tra il termine per la presentazione della richiesta e il termine per il rilascio dell'autorizzazione in proroga costituiscono un intervallo del tutto incompatibile con qualsiasi possibilità di valutare nel merito 5.300 è una proroga generalizzata e indifferenziata a tutte le discariche di rifiuti inerti

tende a valorizzare quanto è già di fatto previsto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 che tratta una materia molto delicata e importante.

Questo emendamento è stato ritirato, come altri del relatore, nella considerazione che il Governo in sede di approvazione e di discussione della legge comunitaria ha aggiunto un *addendum* alle direttive da recepire, che è stato già accolto sotto forma di emendamento dalla 14a Commissione. Mi è ghiotta l'occasione per sollecitare il Governo, dal momento che in quell*'addendum* questa è sicuramente la direttiva più urgente da

il contenuto dell'emendamento del senatore Barelli corrisponde perfettamente all'attuale disposizione di norma esistente nel nostro ordinamento. Vi sono state alcune circolari emanate dal Ministero che hanno indotto in errore anche organi di polizia giudiziaria e organi della magistratura. L'invito al ritiro rivolto al senatore Barelli, quindi, è ispirato ad una correttezza nell'impianto normativo, per evitare ripetizioni o norme interpretative di norme che sono assolutamente chiare; unisco quello al Governo di evitare in maniera assoluta che circolari del Ministero possano derogare a norme di legge. Le leggi le fa il Parlamento, non le fanno i Ministeri con le loro circolari.

anche se sotto forma di possibilità, al regime della TIA, quindi se il senatore Fluttero volesse trasformarlo in ordine del giorno potrebbe essere utilizzato poi o dal Governo o dal Parlamento in una revisione strutturale dell'argomento TIA.

Il Governo è sostanzialmente d'accordo con quanto ha espresso il relatore, ma farà comunque alcune puntualizzazioni.

l'emendamento 5.2, facendo però osservare al presidente D'Alì che la vacanza si verifica solo fino al 31 giugno 2009,

Questa è mancanza di rispetto. Prego, senatrice Mazzuconi.

perché le forme associative volontarie spesso riguardano i consorzi enti parco. Diventava perciò difficile per i Comuni procedere alla creazione di nuovi soggetti,

a tener conto delle valutazioni sopra illustrate, consentendo ai Comuni, nella definizione della tariffa TIA, per le sole utenze domestiche di adottare il criterio pro capite,

una somma da destinare al sostegno dei cittadini in difficoltà economica, assegnabile tramite l'utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. ci tenevo a leggere questo testo perché è una formulazione che abbiamo condiviso all'unanimità in Commissione e ci farebbe piacere che il Governo potesse accoglierlo.

accolto dal Governo, non

Coronella, e che riguarda un tema di cui il Parlamento nelle Commissioni ambiente di Camera e Senato si è occupato: si tratta del decreto legislativo che recepisce la direttiva sulla raccolta delle pile. Per essere molto sintetico, in quella occasione, malgrado un parere unanime espresso dalle Commissioni ambiente sia del Senato che della Camera, sul testo che ci era stato trasmesso dal Governo, il testo poi licenziato dal Governo stesso non solo non ha tenuto minimamente conto del parere delle Commissioni, ma era anche sensibilmente difforme dal testo che ci era stato presentato per il parere. Attraverso questo emendamento cerchiamo di di ribadire un rapporto di correttezza, di fiducia e di lealtà tra il Governo e le Commissioni, in questo caso parlamentari, e nel merito cerchiamo di creare le condizioni perché il tema della raccolta delle pile e soprattutto il tema legato al ruolo del consorzio per le batterie esauste, che in Italia è un organismo che ha dato risultati straordinari dal punto di vista quantitativo e qualitativo un'esperienza di eccellenza invidiata in tutta Europa), non vengano dispersi ed azzerati come sarebbe sulla base del testo del decreto legislativo così come uscito dal Consiglio dei ministri. il Governo voglia accedere a questo emendamento che ha lo scopo di dare il tempo necessario al Governo stesso di ritornare su quel testo e modificarlo in un senso più rispondente alle osservazioni che le Commissioni parlamentari

Come sapete, questa norma derivava proprio da una direttiva europea che ci chiedeva l'apertura al mercato e la fine di fatto della condizione di monopolio

legato all'Unione europea, però l'articolo 6 contiene una proroga che rischia di ributtarci di nuovo

che la norma precedente era nata per ovviare a un problema legato a una procedura europea di infrazione. Con questa proroga, ci rimettiamo dunque in condizioni di assoluta difficoltà quando non di inadempienza.

Ho constatato che ci sono alcuni emendamenti, anche del relatore ed anche approvati in Commissione, che poi sono stati dichiarati in questo consesso inammissibili per diverse ragioni

che gli Stati membri non sono certo tenuti ad adeguarsi prima che vi sia il termine perentorio, ma in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall'adottare disposizioni

l'ideale non è quello di andare avanti con gli emendamenti, ma di procedere ad una revisione organica con una legge, e siccome ci sono già diversi disegni di legge depositati sia alla Camera che al Senato, ci saremmo aspettati un'idea complessiva,

del regolamento e della normativa comunitaria. Quindi, mi aspetto che lei mi rassicuri in questo momento, signor Sottosegretario, sul fatto che tutto ciò che noi stiamo approvando in questo consesso sia in piena sintonia con tale regolamento, per evitare che la Corte di giustizia, anche sollecitata da interessi privati legittimi, possa annullare il lavoro che noi stiamo facendo e aprire eventuali procedure

all'esigenza di molte imprese che, in questa fase difficile di crisi, hanno il problema di non potere detenere nei loro magazzini, di non poter stoccare le cosiddette materie prime secondarie,

Ho una riformulazione da sottoporre al Governo e quindi chiederei l'accantonamento di

riguarda il tema della riduzione dei rifiuti, ma se lo limitiamo al fatto che gli enti locali possono individuare appositi spazi pubblici in cui svolgere periodicamente il mercato dell'usato, diciamo una cosa che è già possibile. Certo, c'è tutta la parte degli accordi, che è aggiuntiva ed utile. Tuttavia accade che nelle aree più virtuose del nostro Paese

di beni ancora funzionanti. Questo però si scontra con il fatto che se questi beni rientrano nell'ambito della raccolta differenziata, non appena entrano in un impianto, qualunque esso sia, ivi comprese le piattaforme autorizzate,

consentirebbe alle associazioni già regolarmente coinvolte nell'ambito della raccolta differenziata - parlo quindi di associazioni *non profit*, ma che hanno tutte le autorizzazioni previste anche per il trasporto e la lavorazione dei rifiuti

raccolta differenziata, a condizione che i beni che entrano nelle piattaforme non si vedano applicato il codice del catalogo europeo dei rifiuti

Pertanto, lo stoccaggio di beni usati funzionanti che possono essere usati per la vendita e ai quali non verrebbe applicato il codice CER,

propongo l'istituzione di un apposito registro. Questo concorrerebbe alla riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento e consiglierebbe il riutilizzo, anche sociale,

al Governo l'accoglimento degli emendamenti 7.0.6/2 e 7.0.6/3 (testo 2), perché per le aree virtuose del nostro Paese questo concorrerebbe davvero ad organizzare meglio le raccolte e gli smaltimenti e comporterebbe una riduzione dei rifiuti avviati avviati definitivamente a smaltimento, sia i rifiuti ingombranti, sia i rifiuti di altro tipo.

Li ritiro, Presidente.

Onorevoli colleghi, come convenuto ieri sera dalla Conferenza dei Capigruppo, nella seduta antimeridiana di domani saranno posti all'ordine del giorno il seguito della discussione del decreto-legge in materia ambientale e i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In ogni caso, anche ove non concluso il decreto-legge, saranno discusse le relazioni della Giunta che rivestono carattere di urgenza. La seduta pomeridiana di domani non avrà luogo. **Interpellanze